L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per i beni e le attività culturali.

Grazie Signor Ministro, con il decreto legge n. 201 del 2011 è stata tolta la competenza alle Regioni sulle decisioni relative alle aperture degli esercizi commerciali. Le attività produttive sono una materia che ha bisogno di essere delegata alle Regioni. Vi sono necessità diverse legate anche alle condizioni climatiche, ai costumi locali, alle zone metropolitane, ai centri turistici, alle zone periferiche, nonché ai Comuni di confine. Lei stessa, lo scorso 29 maggio, ha presentato come prima firmataria un disegno di legge che interviene sulla materia. Nella relazione introduttiva si fa riferimento alla possibilità di attribuire nuovamente alle Regioni la competenza normativa sugli orari di vendita. Dopo il decreto-legge del 2011 si è assistito infatti al fiorire di grandi centri commerciali. Potendo lavorare in condizioni economiche assai differenti hanno portato alla chiusura di piccoli negozi, impossibilitati a garantire l'apertura domenicale. Sulla base di queste considerazioni, le chiedo di sapere se non ritenga che, in sede di revisione della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, in relazione alla quale sono attualmente all'esame della Camera diverse proposte di legge, non sarebbe opportuno riportare nell'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome le decisioni relative alle aperture degli esercizi commerciali.

Nella domanda che viene posta viene chiesta un'opinione in merito a un certo tipo di trattamento e disciplina, quella che riguarda gli aperture domenicali.

nel concreto gli orari di apertura anche in relazione alle loro esigenze territoriali. Trattandosi quindi di una questione che viene trattata in Commissione, ci sarà un dibattito in tale sede

dell'occupazione. Le destinazioni balneari sono le preferite dal 68 per cento dei turisti, che si dichiarano molto soddisfatti dei servizi offerti, con ben 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti nel settore. Signor Ministro, evito i riferimenti normativi, perché penso li abbia già letti nell'interrogazione. Vorrei soffermarmi su alcuni punti a me cari. Lungo tutta la nostra penisola gli stabilimenti balneari rappresentano un comparto economico fondamentale che non può essere lasciato in balia di una normativa ancora incerta. Occorre una legge di riforma che dia garanzia a queste imprese e che tuteli le specificità della loro attività. Nel corso degli ultimi decenni gli operatori balneari hanno migliorato, con il proprio lavoro, sacrifici e investimenti, l'aspetto e la funzionalità delle nostre coste, fino a renderle il simbolo dell'eccellenza turistica che il mondo ci invidia. Questo patrimonio, che non è soltanto economico, ma culturale e direi addirittura identitario del nostro Paese rischia di essere svilito come una qualsiasi merce senz'anima. nostro dovere evitare che ciò accada, tutelando le migliaia di piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno dato vita e corpo al settore, sottraendole alla speculazione delle multinazionali. I Governi che si sono succeduti - nessuno escluso - in questi anni hanno manifestato, soprattutto attraverso l'impugnativa delle leggi regionali, una visione molto parziale dei principi comunitari, invocando esclusivamente l'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein e l'obbligo di trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione dei beni pubblici, trascurando però del tutto due altri principi fondamentali: la tutela della certezza del diritto e la tutela della buona fede di chi ha confidato in un assetto normativo e amministrativo previgente. Alla luce di tutto ciò, tutto ciò, vorrei chiedere al Ministro qual è l'intendimento del Governo per salvaguardare questo importante settore economico del Paese; se non ritenga di valutare l'opzione di rinunciare all'impugnativa proposta dal Governo *pro tempore* Gentiloni e se non ritenga che la rinuncia al ricorso costituirebbe un importante atto politico del Governo a concreta conferma di un'inversione di tendenza rispetto ai Governi precedenti. Allora sì, potreste dare un primo concreto segnale di rappresentare il Governo del cambiamento che rivendicate di essere.

Tra l'altro, le leggi regionali che voi citate cercano di andare incontro a delle esigenze concrete che sono decisamente meritevoli di una seria attenzione, per i motivi peraltro esposti nell'atto di

rinnovo. Noi sappiamo che - purtroppo - la disciplina delle concessioni demaniali è stata già oggetto di una procedura di infrazione avviata e chiusa con il recepimento della tanto contestata e discussa direttiva Bolkestein. Conosciamo bene i commenti che ci sono stati in merito

di analizzare e trovare la soluzione più adatta per affrontare e risolvere la questione a livello normativo, proprio con riferimento al recepimento della direttiva.

intervenire in replica la senatrice Ronzulli, per due minuti. non ci soddisfa, anche perché, alla luce della mozione presentata proprio in quest'Aula il 27 giugno, il Governo si era impegnato ad uscire dalla direttiva Bolkestein.

Comunque purtroppo, come dicevo, la sua risposta non solo non ci soddisfa, ma ci spaventa; penso d'interpretare il sentimento di molte famiglie italiane, che in questo momento stanno ascoltando anche in diretta Grazie

la situazione di migliaia di famiglie, che da anni vanno bussando alle porte di qualsiasi partito. In questo caso, infatti, stiamo parlando di una cosa trasversale, che sarebbe andata aiutare tantissime famiglie. Con questa decisione vi prendete oggi la responsabilità di non aver risolto il problema.

Ieri ha avuto luogo un passaggio importante e assolutamente non scontato (personalmente non ci avrei scommesso): il Parlamento europeo è riuscito a trovare un punto di equilibrio importante - dopo aver rinviato

anche cercando di differenziare il guadagno e le entrate dei grandi gruppi economici che si muovono nella rete dall'attività dei semplici cittadini e dei piccoli *blog* e gruppi d'informazione, che vengono completamente esclusi

con questa direttiva e con tutte le norme sul diritto d'autore è che, se qualcuno ci guadagna (e qualcuno ci guadagna anche molto), quei guadagni vengano redistribuiti e arrivino soprattutto a chi ha davvero lavorato, con la propria mente e con la propria creatività. Questo è il contenuto della direttiva, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo sentito in queste ore, purtroppo anche da colleghi di Governo - a partire dal Vice Presidente del Consiglio passando per alcuni Sottosegretari, che purtroppo hanno la delega in questa materia - che hanno parlato di censura, di un intervento che blocca la rete e che la chiude. Ci domandiamo allora anche perché e quali interessi si vogliono tutelare; perché bisogna scegliere, signor Ministro. Ci sono grandi *player*, i grandi i grandi giocatori dell'economia digitale che vogliono, comprensibilmente dal loro punto di vista, fare i loro interessi senza avere nessuna regola, in una

per capacità di entrate rispetto al diritto d'autore, per le quali vantiamo, ad esempio, nei confronti degli Stati Uniti

che debba essere molto chiaro che cosa vuole fare questo Governo; credo che se ne debba prendere carico fino in fondo il suo Ministero e credo che bisogna combattere qualsiasi tentazione, compresa quella di chi dentro la Rete vuole mantenere il *far west*, perché in tale condizione prospera. Ecco, noi crediamo che sia venuto il tempo di mettere le regole nella Rete, perché le regole garantiscono la libertà, non la tolgono; le regole sono l'unico modo di garantire davvero la libertà per tutti e non il *far west*

Signor Presidente, ringrazio il senatore Rampi per questa interrogazione che mi consente di fare un breve ragionamento sul tema del *copyright* e sugli effetti della direttiva.

proseguirà il proprio *iter* legislativo con i negoziati e, come giustamente dice il senatore interrogante, ci sarà un intervento del Governo, insieme alla Commissione, per far sì che la cosa vada nella direzione giusta. Inizierei ricordando e precisando che non si intende in alcun modo negare la rilevanza del diritto d'autore e del riconoscimento di un adeguato livello di protezione e tutela per gli autori, che è fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell'industria creativa. Il diritto d'autore è infatti fondamentale per assicurare che i creativi e chi lavora in questa industria abbia un'equa remunerazione del proprio ingegno e della propria creatività. Tuttavia, non si può non rilevare che la direttiva in discussione non sembra costituire uno strumento adeguatamente ponderato che coniuga i principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza in modo da fornire un equo bilanciamento tra la tutela del diritto d'autore e la libertà, costituzionalmente sancita, di espressione sulla rete Internet, mostrando un netto e innegabile squilibrio a favore del primo. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 11 che introduce il diritto degli editori di autorizzare o bloccare l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni e l'obbligo di remunerazione a favore di questi per la condivisione anche solo degli *snippet*, che sono le brevi, se non brevissime, anticipazioni degli estratti degli articoli; e all'articolo 13, sui contenuti che i cittadini vogliono condividere e di cui si bloccherebbe il caricamento. Questa è una gravissima imposizione, anche economica, per gli operatori e soprattutto porterebbe alla censura, spesso immotivata, o per la presenza di minime parti di opere, il rischio che intervenga, anche nei casi di utilizzo consentito delle opere, il cosiddetto *chilling effect*, che sarà esponenzialmente incrementato se la nuova direttiva dovesse entrare in vigore. I rischi derivanti dalla direttiva non afferiscono solo alla libertà di espressione e comunicazione, ma anche soprattutto alla limitazione del pluralismo informativo e della libertà di reperire più fonti di informazione. In conclusione, dunque, la mia valutazione, in linea con quella espressa dal vice presidente Di Maio, è negativa e il Governo continuerà il proprio impegno a tutela della libertà e dell'indipendenza della rete, a beneficio della collettività e dei cittadini. La ringrazio ancora per la domanda.

a costruire questo equilibrio. Però bisogna fare una scelta: essendo stati esclusi i *blog* e ad esempio le piccole piattaforme, è evidente che la libertà d'espressione e il pluralismo sono garantiti. viene chiesto con questa normativa è di garantire il fatto che i grandi gruppi agiscano correttamente per distribuire le risorse e lo facciano davvero facendosene carico, perché oggi in linea teorica i divieti c'erano già, ma se nessuno è responsabile nessuno li applica. Pertanto su questo le chiediamo un ripensamento, che c'è stato anche su altre questioni, e le chiediamo un approfondimento che potremmo fare magari anche insieme alle Commissioni parlamentari. Prendiamo seriamente questo tema perché ne va veramente della

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, intervengo per la prima volta in quest'Aula e non posso nascondere l'emozione. Spero mi perdonerete, quindi, se ho scelto di leggere un quesito che, da archeologa che collabora da un ventennio con il Ministero per i beni e le attività La domanda che le pongo, signor Ministro, trae spunto dalla situazione odierna della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (SABAP) per la città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, che dal 2015 al 2018 ha cambiato dirigente ben dieci volte. Avocazioni del direttore generale, reggenze affidate a soprintendenti di altre Province o Regioni, ricorso al cosiddetto comma 6 sono espedienti utilizzati in ogni parte d'Italia, quando occorre; il record raggiunto dalla più meridionale delle due SABAP calabresi, però, difficilmente potrà essere eguagliato. Sottolineo questo infelice primato della mia Regione, mentre auspico che non sia incrementato ulteriormente. Vengo perciò a chiederle se, avendo dichiarato di voler affrontare l'annoso problema della carenza di organico che affligge il suo Ministero a tutti i livelli, diventata ormai intollerabile, vorrà adoperarsi per assicurare anche un congruo aumento del numero dei soprintendenti. Come sa, sono trascorsi oltre dieci anni dall'ultimo concorso, perciò anche le graduatorie degli idonei (dopo quelle dei vincitori) sono state esaurite. Negli archivi le cose non vanno meglio, a quanto mi consta, anzi la situazione è forse addirittura più drammatica. Tuttavia, tornando alle Soprintendenze, Regioni come Calabria, Basilicata, Molise e con esse molte Province (Benevento e Caserta, per fare degli esempi) geograficamente o mentalmente periferiche rispetto ad un MIBAC romanocentrico per tradizione, scontano anche il fatto di non essere scelte come sedi se non dai residenti e solo a condizione che questi non abbiano ambizioni di carriera. Al Sud, infatti, gli interpelli di dirigenti e funzionari che finiscono deserti sono da tempo la norma, dovendo costoro fare i conti con gravi disagi di ordine logistico non compensati né da incentivi economici né da vantaggi di carriera. Per restare all'esempio iniziale, i soli dirigenti, tra quei dieci, passati fugacemente per Reggio Calabria e Vibo Valentia negli ultimi tre anni, o erano ad un passo dal pensionamento o sono stati persuasi ad accettare l'incarico nella prospettiva di risalire la Penisola al più presto per occupare sedi più gradite. Nei casi peggiori - e in Calabria abbiamo visto anche questo la scelta controcorrente di un dirigente nasconde l'esilio dorato al quale personaggi scomodi o imbarazzanti si sottomettono di buon grado per sottrarsi all'attenzione dei superiori. È intuitivo che tutto ciò penalizza enormemente territori ricchissimi sul piano della quantità e della qualità del patrimonio culturale; non di rado questi sono pure vulnerabili agli appetiti di consorterie mosse da interessi economici milionari, risoluti ad approfittare della resa senza condizioni cui l'improvvida riforma Franceschini ha condannato gli ormai anacronistici paladini della tutela. È anche un problema di risorse, infatti, quello che pongo. Perciò, signor Ministro, sempre in relazione alla necessità di aumentare il numero dei soprintendenti, e in attesa che dalla natura trinitaria riconosciuta loro dal suo predecessore ritornino felicemente "monofisiti", le chiedo se non intenda cercare di reperire nuove risorse per assicurare la copertura economica di quei posti di seconda fascia che sono stati penalizzati per pagare stipendi di prima fascia alla folla dei direttori dei musei autonomi, generata anch'essa dalla riforma a costo zero e uguale risultato imposta dal precedente Esecutivo. La

il processo di riorganizzazione del Ministero ha comportato l'adozione di misure di ristrutturazione e razionalizzazione organizzativa, che però non hanno portato gli effetti sperati a causa della grave mancanza di personale. Purtroppo questa situazione non è stata risolta, se non se non in minima parte, dalle assunzioni effettuate negli ultimi anni con concorso per personale non dirigenziale a scorrimento delle graduatorie, autorizzato in deroga al blocco del *turn-over* in occasione di eventi straordinari come sisma e piani di sicurezza. Di questo ho già parlato in diverse occasioni, per cui in questa sede cercherò di essere un po' più analitico, condividendo con voi alcune cifre. In questo momento il Ministero registra un *deficit*, rispetto all'attuale pianta organica di 3.260 unità (siamo circa 16.000), di cui 23 dirigenti. Questa carenza rischia, purtroppo, di aggravarsi nei prossimi anni. In una proiezione che abbiamo svolto internamente, sulla base della cessazione dal servizio prevista tenuto conto dell'età anagrafica dei dipendenti, evidenzia che nel triennio 2019-2021 il *deficit* di personale salirà a 4.431 unità, di cui 39 dirigenti, mentre nel 2022-2024 crescerà ulteriormente per arrivare a 7.893 unità, di cui 66 dirigenti. Questa, purtroppo, è una stima prudenziale che sto facendo in base alle attuali regole di collocamento in pensione; pertanto, nel momento in cui si dovesse riformare la legge Fornero, questi numeri potrebbero aumentare anche in maniera significativa. Il Ministero ha messo in atto, in primo luogo - e qui rispondo alla richiesta di informazioni sulla mancata assunzione di dirigenti negli ultimi anni - alcune misure urgenti immediate, volte al reclutamento di personale dirigenziale. Nel mese di luglio abbiamo richiesta al Ministero della funzione pubblica l'autorizzazione a bandire un concorso per la selezione di cinque dirigenti architetto e quattro dirigenti archeologi. Nel mese di agosto il Ministero ha chiesto di essere autorizzato ulteriormente a bandire un concorso per 17 dirigenti tecnici (archivisti e amministrativi) e ad assumerne altri 9 (storici dell'arte) con scorrimento della graduatoria. Nella stessa ottica, a luglio, abbiamo sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo per l'espletamento di un concorso interno per il passaggio di area del personale in servizio. Infine, il Ministero sta collaborando attivamente con il Ministero della funzione pubblica per un piano straordinario volto al reclutamento del personale dirigenziale e non. In particolare, nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno, abbiamo inoltrato al Ministero della funzione pubblica la richiesta di bandire un concorso per l'assunzione di un totale di 4.377 unità, di cui 2.943 di area II e 1.434 di area Abbiamo inoltre rappresentato l'intenzione di assumere 39 dirigenti mediante scorrimento delle graduatorie, in modo da coprire interamente il fabbisogno dirigenziale che nelle more si sarà determinato per effetto della cessazione dal servizio. È mia intenzione, al momento di indire i concorsi, individuare un ordine di priorità dei profili ritenuti più urgenti, sulla base delle indicazioni che ho raccolto, in particolare proprio dalle Soprintendenze. Anche di recente, la scorsa settimana, ci siamo trovati al Ministero e, alla presenza di tutti i soprintendenti, abbiamo raccolto le loro indicazioni. La ringrazio ancora intervenire in replica la senatrice Corrado, per due minuti. *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio. Mi ritengo soddisfatta. Aggiungo soltanto l'auspicio di tornare al più presto a livelli occupazionali adeguati all'importanza del suo Ministero, destinando alla cultura le risorse che merita in un Paese come il nostro.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario dei lavori in relazione alla prevista terza lettura del decreto-legge recante proroga di termini legislativi, tuttora all'esame della Camera dei deputati. Nella giornata di martedì 18 settembre l'Assemblea non terrà seduta

Nella seduta di mercoledì, che non prevede orario di chiusura, si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale. I tempi di esame sono stati rimodulati in base a specifiche richieste dei Gruppi. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 19. Resta confermato alle ore 15 di giovedì 20 lo svolgimento del *question time*. Infine, nella seduta di martedì 2 2 ottobre, alle ore 17, il Ministro degli affari esteri renderà la prevista informativa sugli sviluppi della situazione in Libia.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Basilicata si vive una condizione di disastro ambientale con gravi rischi per il territorio e per la salute umana, come ben sa anche il ministro dell'ambiente, Sergio Costa, dato che il suo primo viaggio istituzionale l'ha riservato proprio alla Basilicata. In questa Regione ci sono due aree SIN di bonifica nazionale, Tito e Pisticci Scalo; sono state realizzate ben 474 perforazioni tra pozzi attivi, sterili ed esausti (mi riferisco all'annosa questione del petrolio); si cerca petrolio fino a 4 chilometri di profondità, con enormi costi ed enormi rischi sul sistema idrico del sottosuolo lucano; esistono tre centri oli, dei quali uno, quello di Viggiano, grande ben 18 ettari, è al centro di gravi polemiche per la sua vicinanza a uno dei bacini idrici più grandi della Basilicata, il Pertusillo. Questo centro oli ha una rete di oleodotti di ben 750 chilometri che attraversano un delicatissimo bacino idrico molto importante, quello del fiume Agri, che oltre all'invaso del Pertusillo, ha 650 sorgenti di acqua purissima che producono 3.000 litri al secondo di acqua potabile. Ci sono poi nel nostro Paese ben 44 discariche non a norma, che sono state motivo di recente deferimento dell'Italia da parte della Commissione europea, ben 23 delle quali si trovano in Basilicata. Inoltre, nell'area più produttiva della Basilicata, il Metapontino, per l'agricoltura di qualità e un turismo diffuso, che tra l'altro è area di bonifica europea per i nitrati, oramai si vive in costante emergenza di trialometani, periodicamente presenti nel circuito dell'acqua potabile. Nell'area di Melfi esiste un vecchio inceneritore, la Fenice, che brucia 35.000 tonnellate di rifiuti industriali più 30.000 tonnellate di rifiuti urbani. Nel 2011 furono arrestati il direttore generale e un dirigente dell'ARPAB, in relazione ai dati di inquinamento delle falde idriche sotto l'inceneritore di Melfi tenuti nascosti per ben nove anni. Secondo la procura di Potenza, ed è cronaca recente, attorno all'inceneritore di Melfi c'è stata «la diffusione di inquinanti all'esterno» della struttura, con la «compromissione delle acque potabili e grave pericolo per la salute pubblica». In virtù di ciò, il

questa lunga premessa per portare un grido di aiuto dalla Regione Basilicata in quest'Aula, per chiedere un intervento diretto, visti i reiterati insulti all'ambiente da almeno un decennio procurati da questo catafalco di inceneritore, arrivando ad ordinarne la chiusura definitiva per i reiterati rischi procurati all'ambiente. Tutto Tutto questo perché oramai, grazie anche alla cronaca e alle azioni della procura, oggi sappiamo che almeno per le contaminazioni delle falde idriche dell'area del Vulture abbiamo un colpevole conclamato: l'inceneritore di Melfi. A questo punto bisogna assolutamente chiuderlo, una volta per tutte, a tutela della salute pubblica delle persone. *(Applausi